e soprattutto di rispetto reciproco, che si sta tenendo in Commissione ci faccia perdere di vista il fatto che ci troviamo di fronte a una richiesta, l'ennesima, di rinvio dei lavori. Come si sa, alla fine dell'anno precedente, dopo le gravi violazioni dell'articolo 72 della Costituzione nell'*iter* di approvazione della legge di bilancio, il Gruppo del Partito Democratico ha sollevato il conflitto di attribuzione presso la Corte costituzionale.

perché non ci sono le condizioni per sviluppare un ragionamento di merito che vada nella direzione di sciogliere un dubbio politico, che - con ritardo e confusione - viene sciolto esclusivamente dal Governo. Peccato che, per l'ennesima volta, questo accada

alla procedura, dobbiamo riconoscere alla maggioranza e al Governo un cambio di passo. In Commissione stiamo lavorando in maniera costante e continuativa. Abbiamo avuto l'impegno, da parte dei Presidenti delle due Commissioni di merito, del Capogruppo

ci sono molte cose da dire, e le diremo nel corso dell'esame del provvedimento, dobbiamo prendere atto con onestà intellettuale che quantomeno da questo momento comincia un'inversione di tendenza, con un maggiore rispetto delle funzioni parlamentari e quindi anche di quelle che devono svolgere i rappresentanti dell'opposizione.

un approfondimento e di dare un contributo da parte delle Commissioni. Solo in questo modo, infatti, si ripristina il regolare andamento dei lavori e la centralità delle Commissioni del Parlamento.

riferito dal presidente Coltorti, non possiamo che sospendere la seduta. Avverto che la Conferenza dei Capigruppo si riunirà alle ore 10,

nelle sedute di giovedì 24 e, ove necessario, venerdì 25. Le sedute non prevedono orario di chiusura. La relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia sarà anticipata alle ore 9,30 di domani, secondo i tempi già definiti. Il sindacato ispettivo

in particolare il motivo per il quale siamo usciti non con un verdetto unanime, bensì a maggioranza. Anche oggi il collega Vitali ha sottolineato alcuni aspetti del lavoro di Commissione sul decreto-legge semplificazioni, che rischia di diventare uno dei provvedimenti più complessi ed eterogenei della storia di questa legislatura. Per noi non c'è stato alcun intento e non abbiamo manifestato alcun atteggiamento ostruzionistico. Con i nostri emendamenti

ampiamente allargato il perimetro di applicazione del decreto-legge semplificazioni, rendendolo di difficilissima applicazione ed è proprio su questi temi che abbiamo perso tempo. È semplice e molto complicato

la difficoltà, lo stato confusionale, la profonda difficoltà di interazione tra le due componenti della maggioranza. Di questo, però, non possiamo essere accusati noi e non possiamo nemmeno ogni settimana ritrovarci qui a dire che alla fine ne subiamo le conseguenze, ne subiamo le conseguenze, perché il calendario di quest'Assemblea cambia. Per quanto riguarda noi, *nulla quaestio* nell'invertire l'ordine dei fattori

Va bene cominciare a esaminare il decreto-legge semplificazioni in tutta la sua complessità domani pomeriggio; va bene utilizzare tutta la giornata di giovedì per lavorare sul decreto-legge semplificazioni.

il ministro Moavero per sapere che intenzioni ha o se ha un parere, una posizione omologa, lievemente diversa o totalmente dissonante rispetto alle dichiarazioni rese dal ministro Di Maio. Tutto questo però, visto che la maggioranza ha mancato il suo patto nei confronti delle opposizioni, rende molto difficile combinare il calendario. Capite quante conseguenze ha la continua rottura del patto di lealtà parlamentare della maggioranza nei confronti delle opposizioni: ogni volta deve cambiare qualcosa. *(Applausi dal Gruppo una seduta nella giornata di venerdì, naturalmente compatibilmente con la disponibilità del ministro Moavero, per capire che ne sarà noi e dei nostri rapporti con la Francia. Su questo siamo d'accordo, ma, signor Presidente, vogliamo - e con questo concludo e chiedo ai colleghi ancora un attimo di pazienza - che finalmente si applichi il Regolamento del Senato come è stato modificato di comune accordo la scorsa legislatura, creando un'alternanza operativa tra il lavoro dell'Assemblea e quello delle Commissioni, cosa che non è ancora avvenuta. Chiediamo quindi che sia confermato il calendario della prossima settimana, che vede lavorare solo le Commissioni, che non ci siano contaminazioni di sorta e chiediamo con forza alle componenti di sorta e chiediamo con forza alle componenti della maggioranza che nulla cambi di quello che è stato per l'ennesima volta rinegoziato tra la maggioranza e le opposizioni stesse. Ribadiamo naturalmente la nostra richiesta di calendarizzazione delle mozioni. alla mozione di cui ho parlato la scorsa settimana sul monito del Presidente della Repubblica e sulla conseguente deliberazione della Corte costituzionale, che apre nuovi spaccati sul ruolo di tutti noi; alla mozione sull'autismo e sulle gravi disabilità;

Signor Presidente, esprimo la contrarietà del Gruppo Partito Democratico al calendario così come presentato senza

un mezzo sfondava addirittura il portone di un Ministero. Mi chiedo, se in Italia in questo momento sfondassero il portone del Ministero dello sviluppo economico,

Ci sarà certo occasione di approfondire questi temi quando il ministro Moavero ci farà la cortesia di venire in Aula, che stiamo assistendo a un cambio radicale della politica estera del nostro Paese, che tradisce di fatto i nostri interessi nazionali. Quando c'è da discutere in Europa delle modifiche al nuovo piano pluriennale per assegnare le risorse, il quale vede dare molti meno soldi nell'ambito della politica agricola comune agli agricoltori italiani e abbiamo la possibilità di recuperare solo alleandoci con la Francia, non si tratta di interesse nazionale? Ci inimichiamo il principale *partner* in Europa che ci può aiutare a recuperare risorse? E lo stesso vale per l'allentamento dell'*austerity*. Chi in questo momento in Europa ha i nostri stessi interessi nell'allentare le regole europee? Chi è tra i commissari quello che ha guardato con più favore a non aprire la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia se non il commissario francese?

assolutamente sereno. Quindi, meglio un giorno in più di dibattito che l'assenza di dibattito, come colpevolmente il Governo aveva imposto al Parlamento in occasione della legge di bilancio.

alla richiesta di ascoltare il ministro degli affari esteri Moavero. E credo sia favorevole, senza

la decisa presa di posizione contro certi atteggiamenti neocolonialisti della Francia. Voglio evidenziare - non è una gara alla primogenitura, ma basta guardare sul *web* - che Fratelli d'Italia per primo, insistentemente, con Giorgia Meloni, sin dalla nostra manifestazione di settembre «Atreju», ha cercato di far entrare il tema nel dibattito politico. Non possiamo che essere contenti quando le nostre tesi appaiono sulle labbra dei nostri avversari politici, quali sono i componenti del Governo di cui non facciamo parte. Mi rivolgo agli amici del PD: capisco la vostra strenua difesa

un effetto di copertura di numerosi terroristi presenti in Francia. Avete difeso - e non lo dimentico - i sorrisini di Sarkozy con la Merkel, quando si prendeva in giro l'Italia. *(Applausi dai Gruppi

dai *gilet* gialli che lo stanno sbeffeggiando in Francia. Capisco ed è legittima la posizione della sinistra in difesa della Francia; meno legittimo è lo stravolgimento di una posizione politica, per noi assolutamente negativa, che vede da sempre la Francia non concorrere alla possibilità di fare dell'immigrazione un evento in qualche modo gestibile. Siamo assolutamente convinti che l'immigrazione non sia bloccabile, ma debba essere gestita. La Francia ha contribuito a rendere all'Italia ingestibile o difficilmente gestibile la questione dell'immigrazione, per quanto attiene alle nostre frontiere, e ha altresì contribuito a rendere l'Africa un luogo dal quale è più facile scappare piuttosto che cercare di rimanere e costruire qualcosa. Per questo motivo ascolteremo con piacere quanto il ministro Moavero, riprendendo le tesi di Fratelli d'Italia e Georgia Meloni, ha intenzione di dire e di fare su detta questione.

Presidente, conosce perfettamente. Di qui nascono molti problemi e a questo dobbiamo aggiungere le questioni e i nodi politici che

centro per rifugiati, che si trova qui alle porte di Roma, a Castelnuovo di Porto, senza avvertire i sindaci e senza conoscere quale sia la destinazione di tutte le persone che si trovano là dentro. Quindi, si continua con una gestione

del Vice *Premier*, di fare un'operazione di distrazione e di indirizzare tutto verso la Francia. Questa è la questione che, francamente, troviamo insopportabile. Credo quindi sia assolutamente necessario che quest'Aula abbia un'informativa su quello che sta accadendo

intervengo per sottolineare che da parte del Gruppo della Lega non vi è, naturalmente, alcuna contrarietà a a convocare in Aula il ministro Moavero Milanesi e ad ascoltarlo in merito alle vicende che sono state evocate da chi mi ha preceduto. L'unica osservazione è che vorremmo evitare che ciò interferisse ulteriormente con l'ordine dei lavori in merito al decreto semplificazioni. C'è anche da aggiungere qualche considerazione. Secondo me ha perfettamente ragione la collega De Petris quando segnala che, forse, più che sui temi che sono finiti, per certi motivi, sulle prime pagine dei giornali e su cui comunque vorrei aggiungere qualche piccolo commento, sarebbe interessante sapere qual è la posizione del Governo - e siamo interessati a sollecitarla - sul tema del nuovo trattato franco-tedesco e, più in generale, sull'atteggiamento dei nostri cugini francesi e dei nostri cugini tedeschi riguardo all'Europa. L'Europa dovrebbe essere un progetto multilaterale ma, in realtà, si articola sempre intorno a questo asse franco-tedesco e attorno a quella che Martin Feldstein, un eminente economista americano, alla fine degli anni Novanta aveva in qualche modo stigmatizzato come la contraddizione fra l'aspirazione francese all'uguaglianza e il desiderio tedesco all'egemonia. Ecco, queste dinamiche continuiamo a vederle in opera e, ad avviso di chi parla, ma con tutta umiltà, voglio segnalare che mi sembrano un po' disfunzionali rispetto ad un ordinato sviluppo del progetto europeo. Esse sono altresì alla base di alcune tensioni che emergono. Io apprezzo molto che, finalmente, il commissario Moscovici abbia riconosciuto, ieri, che le provocazioni squalificano chi le fa. Credo si rivolgesse a se stesso, a quando, il 13 dicembre dello scorso anno, definì la situazione politica europea come caratterizzata dall'avvento di tanti piccoli Mussolini. Reagì il vice *premier* Salvini e fece bene, perché questo spettro del fascismo, evocato in tutte le possibili salse, non contribuiva certo a rasserenare il clima. Quindi, si può discutere dei toni con i quali i problemi vengono sollevati e si può discutere sulla tempistica con i quali vengono sollevati, ma non mi sembra che questo Governo sia in condizioni di poter accettare lezioni di stile da una Commissione europea che ha già dato prova di essere un pochino incontinente nelle sue critiche. *(Applausi dai

è legato all'euro. Di fatto, quindi, vediamo agganciato a noi e alla nostra economia monetaria un pezzo enorme di Africa sub sahariana e al riguardo occorrerebbe articolare alcune riflessioni. Anche su questo punto sarebbe interessante sentire le riflessioni del ministro Moavero e ci associamo senz'altro alla richiesta di chi ha espresso il desiderio di sentirlo,

la proposta è stata formulata nel momento in cui è stata fatta una dichiarazione sul calendario: c'è quindi il diritto, da parte dei senatori che lo richiedano, di svolgere la dichiarazione di voto sulla proposta

ci hanno davvero rassicurato l'interesse, la passione e soprattutto l'apertura della Lega rispetto all'urgenza di questo dibattito. A tale proposito, oltre

in un'ottica di collaborazione, posso aggiornare la mia richiesta alla settimana prossima, per evitare che ci siano distonie. Se esiste una disponibilità per la settimana successiva, posso rimandare la mia

chiarezza. Ad esempio, io credo che anche durante la settimana dedicata alle Commissioni si possa ritagliare uno spazio per ascoltare, per cui le chiederei che la prima votazione, se possibile,

Anche in seguito alla discussione che c'è stata in sede di Capigruppo, noi chiediamo di mettere in votazione una richiesta esplicita, definita e molto semplice e cioè che in questa settimana, considerate le dichiarazioni del vice presidente Di Maio, le dichiarazioni di questa mattina del vice presidente Salvini e, ovviamente, visto che, a questo punto bisogna prendere atto di una modifica della politica estera del nostro Paese, il Ministro degli affari esteri venga a riferire in Parlamento, non specifico al Senato, con urgenza. rispettando gli impegni che abbiamo preso con la maggioranza sul decreto che stiamo discutendo in Commissione, quindi a seguire, il che significa o giovedì sera o venerdì. Per semplicità di votazione noi proponiamo venerdì, in modo che il Ministro, nell'arco della giornata, dirci se e quando vorrà venire. Ovviamente il Parlamento, per il Governo, non è qualcosa di vario ed eventuale, ma dovrebbe essere una priorità, in particolare su questioni così rilevanti.

apprendiamo che il senatore Lannutti si è scusato per le farneticanti dichiarazioni di ieri. Non è tuttavia possibile non stigmatizzare il continuo ricorso - e in queste ultime ore abbiamo assistito ad una vera e propria *escalation*

ha riproposto come fonte - e questo è davvero pazzesco - "Protocolli dei Savi di Sion", che è l'emblema dei falsi alla base dell'antisemitismo. Siamo alla riproposizione dei più violenti e infondati pregiudizi, alla riproposizione di un autentico falso, cioè della *fake news* più foriera di odio e morte nella nostra storia, lo strumento fabbricato e usato per perseguitare ed eliminare in tante parti del mondo le persone di religione ebraica, dai *pogrom* russi fino ai campi di sterminio nazisti. Sa il senatore Lannutti che in Germania i «Protocolli» - ripeto, un documento totalmente falso, creato al solo scopo di alimentare l'odio contro gli ebrei - furono usati dai nazisti come una licenza per il genocidio?

per conoscere e mai dimenticare la storia dell'Olocausto e la tragedia della Shoah. Penso che chi siede in Parlamento e rappresenta le istituzioni non possa farsi portavoce davanti al Paese di messaggi falsi, irresponsabili, pericolosi e discriminatori. Non si può - e mi rivolgo ai colleghi del MoVimento 5 Stelle - guidare l'Italia e contemporaneamente continuare a distruggerla, ad indebolirla, a minare la sua credibilità internazionale a colpi di bufale negazioniste, razziste, antisemite e discriminatorie. L'Italia è un grande Paese che non merita di essere trascinato così in basso, in una gara continua tra voi, forze di Governo, a chi la spara più grossa,

e che ci giudicano per quello che noi diciamo in queste Aule. Vi prego, fermatevi davvero, prima che sia troppo tardi. *(Applausi

Avendo noi avanzato la richiesta di ascoltare il ministro Moavero nella prossima settimana, anche se è la settimana dedicata alle alle riunioni delle Commissioni, probabilmente quella votazione, se avessi avuto la possibilità di intervenire, lei l'avrebbe disposta. Non le chiedo di farlo ora, perché mi rendo conto che non sarebbe corretto, visto che molti colleghi hanno già lasciato

il più presto possibile, secondo il calendario che lei riterrà di modificare, anche sentendo i Capigruppo, e la possibilità di dedicare tempo a questa incombenza del Ministro stesso. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle in risposta all'intervento della senatrice Fedeli, perché pensiamo che su un argomento così delicato ovviamente non ci si debba sottrarre, ma che bisogna anche chiarire alcuni punti, proprio nel rispetto della delicatezza dell'argomento che avete sollevato.

La chiarezza di questa frase e di questi intenti credo non sia fraintendibile. Ciò detto, credo che anche la senatrice Fedeli conosca la storia umana e parlamentare del senatore Lannutti. Lei ha iniziato il suo intervento dando atto che il senatore si è scusato per le parole che ha scritto sul suo *post* e ha anche chiarito il senso del suo errore e ha dichiarato in maniera netta ed incontrovertibile che non è né antisemita, né contrario a qualsiasi tipo di tipo di confessione religiosa. A questo punto, penso che sia doveroso prendere atto di queste scuse e non costruirci un teorema che si estende alla politica del MoVimento 5 Stelle o anche a quello che sarà in futuro, alla manovra finanziaria, alla politica di questo Governo, perché questo, sì, è scorretto intellettualmente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Penso, senatrice Fedeli, che lei conosca la storia del senatore Lannutti e parla la sua vita, perché se una persona

e ogni forma di complottismo, ogni tesi, ogni teoria sconfessata dalla storia. Non è accettabile che sulla base di questa serissima argomentazione si faccia politica contro il Governo e contro il MoVimento 5 Stelle, perché questo non c'entra nulla. *(Commenti del senatore Faraone).* Colleghi, ve lo dico con molta serenità: siamo intervenuti in risposta, era doverosa una risposta, il senatore ha chiarito il suo errore e si è scusato. Credo che su questo capitolo, almeno in quest'Aula, sia doveroso mettere la parola fine.

che altri non l'abbiano fatto. Adesso, addirittura, si viene attaccati perché ci si permette di citare il problema. Questo mi sembra davvero esagerato. Quando si sbaglia, si chiede scusa.

in cui uno Stato sovrano, che ha ottimi rapporti con l'Italia, continua a minacciare lo sterminio totale degli ebrei che si trovano in Israele. Ciò è pericoloso, e lo sarebbe anche se non fosse la settimana in cui ricorre il Giorno della memoria.

il voler strizzare l'occhio a posizioni pericolose e credo che sia il Gruppo... Ringrazio il collega che dimostra il suo convincimento democratico. Credo che il Gruppo MoVimento 5 Stelle

Signor Presidente, abbiamo appreso oggi da notizie di stampa che l'ex collega senatore Stefano Esposito, il prefetto di Torino e il direttore dell'ANSA hanno ricevuto delle minacce, dei proiettili. Il mio intervento è per esprimere solidarietà e chiedo che solidarietà possa essere espressa anche dall'intera erano indirizzati appunto a queste tre autorità: si tratta di quattro buste con proiettili scoperte al centro di smistamento delle Poste di Torino. Quanto è accaduto è raccapricciante, noi condanniamo fermamente questi vili atti di inciviltà e ci auguriamo che gli investigatori possano al più presto fare chiarezza e individuare i responsabili di questi atti incivili. Chiedo nuovamente all'Assemblea di esprimere solidarietà su quanto accaduto.